Onorevoli colleghi, profondamente addolorato, devo dare all'Assemblea una triste notizia. La scorsa notte è venuto a mancare il senatore Questore anziano Romano Comincioli. Il senatore Comincioli è stato componente della nostra Assemblea a partire dalla XIV legislatura, e ha ricoperto l'incarico di senatore Questore dalla XV. I suoi funerali si terranno domani 15 giugno a Milano, presso la Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11. Pertanto, per consentire la partecipazione ai funerali, non si terrà la seduta antimeridiana di domani che è stata condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo). La commemorazione in Aula avrà luogo in una data successiva, alla presenza della famiglia. In segno di cordoglio e vicinanza ai familiari e amici, vi invito a osservare un minuto di raccoglimento.

In conseguenza della scomparsa del senatore Romano Comincioli, autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi sin da ora per procedere alla individuazione del senatore subentrante nel seggio resosi vacante per la Regione Lombardia. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 23 giugno. Come già ricordato, l'Assemblea non terrà seduta nella mattinata di domani per consentire la partecipazione dei senatori ai funerali del compianto senatore Comincioli, Questore anziano del Senato. La seduta pomeridiana di domani, per la quale non è previsto l'orario di chiusura, sarà dedicata al seguito dell'esame del provvedimento anticorruzione fino alla sua conclusione. Nella seduta antimeridiana di giovedì saranno posti all'ordine del giorno gli altri argomenti già previsti in calendario per questa settimana. Per il disegno di legge concernente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato riaperto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di domani. Il calendario della prossima settimana prevede per martedì 21 giugno, con inizio alle ore 16, il dibattito sulla composizione del Governo che sarà introdotto da un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri. La discussione si esaurirà entro la serata di martedì. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame della mozione su una strategia mondiale per il settore alimentare, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e la mozione sulla sicurezza da minaccia cibernetica. Comunico, infine, che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 23 giugno, alle ore 9, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori.

questa ed altre norme uscivano dal testo non perché ritirate o per un ripensamento, ma perché, di fronte al protrarsi dei lavori delle Commissioni parlamentari, sono state inserite in altri

parere favorevole del Governo

a ritirare l'emendamento 5.250, soppressivo dell'articolo 5, in quanto mi risulta che vi sia la disponibilità ad accogliere l'emendamento successivo che, essendo sostitutivo dell'articolo,

dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura conseguenti a un reale esame della situazione delle imprese. Riteniamo che la lista delle imprese amiche non sia sufficiente,

hanno dei problemi, che devono giustamente essere posti all'attenzione, con aggiornamenti continuativi, delle stazioni appaltanti e degli organi amministrativi a ciò deputati.

Signora Presidente, vorrei sottoporre in particolare al Governo, oltre che ai colleghi, la considerazione che l'introduzione di una *white list*, e cioè di un elenco di imprese in determinati settori dell'attività imprenditoriale, debba essere assistita da un'indicazione specifica

dell'obbligo di indicare eventuali mutamenti di assetti interni all'impresa ai fini della

di emanare una norma inapplicabile e assolutamente inutile, tradendo così le buone intenzioni di tutti, che consistono

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.251 (testo 3), 6.4 (testo 2) 10.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'emendamento 4.2 (testo 2), sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

nel comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 70 del 2001, invito tutti i presentatori di emendamenti

di elenchi che non sono del tutto corrispondenti a quello attuale, ma che possono essere tali da mettere in evidenza l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

inapplicabile in concreto, poiché non è specificato chi terrà questi elenchi (se le prefetture o il Ministero dell'interno) e chi deve fare i controlli, preventivi e successivi.

inapplicabile e inutilizzabile, che tradisce le buone intenzioni di tutti i presentatori e di tutti coloro che si sono affannati su questa vicenda. Se vi è qualcosa di analogo nel decreto‑legge, lo esamineremo successivamente e poi andremo a verificare.

di secretazione degli appalti dal piano politico a quello amministrativo è già stata introdotta dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

che contiene norme diverse che riguardano la risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati. la risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati. Comprendendo la ragione che è sottesa alle argomentazioni del Sottosegretario, il mio intento era proprio quello di sostituire l'articolo 6 con 6.250. Diversamente dovrei dire: sopprimere l'articolo e sostituirlo con il 6.250.

e l'emendamento estende la sanzione civilistica ad una serie di reati del tutto eterogenei, di diversa gravità, che interessano beni giuridici non assimilabili. Per tale ragione, il parere

L'Italia continua a crescere poco; anche gli ultimi dati sottolineano che cresciamo un punto di PIL all'anno, meno della metà della media europea. dovuta a bassa competitività. C'entra questo con l'argomento di oggi? Direi proprio di sì, e direi che c'entra molto. In tutte le statistiche internazionali emerge con chiarezza che per l'Italia la presenza di un'elevata corruzione, di estese ramificazioni di economia criminale, di scarsa trasparenza dei processi decisionali pubblici, costituisce una palla al piede per la competitività del sistema Paese. L'ampia letteratura esistente sull'argomento e i dati empirici dimostrano che c'è una correlazione diretta tra presenza di corruzione e difficoltà della crescita: più corruzione c'è, più bassa è la crescita. Si parla molto - e giustamente lo fa il ministro Tremonti - di riforme a costo zero. La lotta alla corruzione è certamente una di queste riforme e va perciò vista come uno specifico strumento di politica economica. è il grande mare dell'economia sommersa (250 miliardi di euro, pari al 17 per cento del PIL); accanto all'economia informale e a quella che sfugge agli obblighi fiscali e contributivi, si sviluppa una economia criminale, con una capacità invasiva dell'economia formale. Sono ambienti in cui i fenomeni corruttivi possono prosperare: 19 miliardi è il fatturato delle ecomafie, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente. La Corte dei conti ha stimato in 50-60 miliardi di euro all'anno il peso della corruzione, definendola nell'ultima relazione del procuratore generale «una tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche di tutti i cittadini». Cosa vedrebbe un investitore internazionale che volesse investire in Italia e cercasse di orientarsi con le statistiche disponibili? La Banca mondiale pubblica un indice nei *Worldwide Governance and Anti-Corruption Indicators*, che colloca l'Italia al sessantottesimo posto mondiale, penultimo dei Paesi dell'area OCSE, con una perdita di 36 posizioni in dieci anni.

l'Italia compare al quarantottesimo posto, avendo perso 21 posizioni in dieci anni. Particolarmente negativi sono gli indicatori relativi ai pilastri istituzioni e corruzione (settantatreesimi), trasparenza (centodiciannovesimi) e favoritismi nelle decisioni pubbliche (centoquindicesimi). Eurobarometro ci colloca al ventunesimo posto su 27 per presenza di corruzione.

Occorre prosciugare le fonti che alimentano la corruzione: riduzione degli oneri burocratici, semplificazione normativa e procedimentale, trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e attività economica, lotta al riciclaggio di denaro sporco, che è il veicolo principale per chiudere il cerchio della corruzione. Molto può essere fatto rendendo pubblici tutti i dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni, con una evidenza dei costi di produzione di servizi ed opere, strutturati per consentire la confrontabilità con le migliori pratiche. In Gran Bretagna, l'esperienza è in campo, e sta dando frutti importanti. però, avete affossato perfino la parte positiva della riforma della pubblica amministrazione che voi stessi avevate impostato. Pensiamo al ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi: è un tempo triplo rispetto alla media europea. Confartigianato ha calcolato in un miliardo di euro l'onere finanziario aggiuntivo per le imprese del comparto. C'è da meravigliarsi se in questo stato di cose si annidino incentivi alla corruzione? Occorrerebbero pertanto un'azione complessiva ed un atteggiamento culturale costante prima della disponibilità di norme repressive. Per tali ragioni, il disegno di legge in esame rischia di essere una occasione persa. Se pure si fa qualche passo in avanti, troppo timido e limitato, se ne fanno molti indietro con altre proposte legislative. Pensiamo all'allarme esplicito lanciato dalla Corte dei conti sugli effetti devastanti per la lotta per la legalità che sarebbero procurati dalla proposta normativa in materia di intercettazioni e durata dei processi, dalla limitazione introdotta all'attività della Corte stessa, dagli effetti disastrosi dello scudo fiscale nel favorire la ripulitura di denaro frutto di attività illecite. In qualche misura la lotta alla corruzione deve diventare una sorta di infrastruttura civile, solida e condivisa. Se ciò non avviene e se l'opinione pubblica percepisce che per tutte le istituzioni questa non è una priorità e, al contrario, si attacca con frequenza il principio di legalità e chi lo difende, è veramente difficile ottenere risultati apprezzabili. Il parere contrario che il Governo continua ad esprimere su tentativi di miglioramento dell'opposizione - come nel caso dell'emendamento in esame - dimostra che purtroppo l'Esecutivo non intende impegnarsi a fondo su questo documento decisivo per la competitività del Paese.

Invito il senatore Segretario a verificare

Se questa proposta è accettata dal Governo, sono d'accordo, altrimenti interverrò nel merito degli emendamenti.

Presidente, lo ripeto per chiarezza alla Presidenza.

Presidente, gli articoli 7 e 8 sono stati ritenuti dalla

7 ed 8 ripropositivi della Carta delle autonomie, in particolare degli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259, già all'esame del Senato. Ed in tal senso, aderendo anche all'orientamento della Commissione bilancio, il Governo è d'accordo a stralciare gli articoli 7 ed 8, ovviamente riproponendo da parte del Governo e anche dei singoli senatori in quella sede gli eventuali emendamenti.

Presidente, il sottosegretario Caliendo ha già risolto il problema;

Gli emendamenti relativi a questi articoli sono importanti poiché sono relativi al controllo di gestione, ai controlli interni e quant'altro.

Signora Presidente, credo che la posizione espressa dalla senatrice Incostante sia quella più confacente alla realtà. Noi abbiamo

volevo chiedere l'accantonamento anche degli articoli 10 e 11, all'esame dei quali siamo arrivati prima di quanto tutti si aspettassero,

fiscale. Quindi, riterrei opportuno lo stralcio dell'articolo 9, visto che il decreto è già all'esame della Commissione bicamerale, ed entro la fine di luglio diventerà legge.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S9.100, le disposizioni di cui all'articolo 9 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (A.S. 2156-*quater*). Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S9.100, le disposizioni di cui all'articolo 9 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Delega al Governo in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (A.S. 2156-*quater*). Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

abbiamo acceduto all'idea di accantonare la discussione degli articoli 10 e 11 sulla base di un'affermazione del senatore Malan, il quale dice di aver predisposto un nuovo emendamento. Noi non siamo a conoscenza del suo contenuto;

dei Valori, è particolarmente complesso in quanto affronta la materia dell'adeguamento del nostro ordinamento alla Convenzione di Strasburgo

alcuni interventi in materia di reati contro la pubblica amministrazione. I due punti più significativi sui quali richiamo l'attenzione sono rappresentati

è il reato di estorsione commesso dal pubblico ufficiale, ma esistono delle forme di concussione per costrizione e le cosiddette concussioni per induzione, ossia quando il concusso paga il prezzo della corruzione dicendo che comunque sarebbe stato indotto non attraverso richieste o minacce, sia pure implicite, ma da un atteggiamento. Sono delle forme che vengono utilizzate per affrancarsi da una possibile accusa di corruzione per cui il corruttore accampa la propria

contro la pubblica amministrazione in materia di corruzione deve consentire la possibilità di sanzionare tutti i pagamenti fatti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Qualora ci sia la richiesta

la condanna fino a cinque anni per i commercianti che non denuncino il pizzo richiesto dai mafiosi. Chiediamo ai commercianti di fare gli eroi (diversamente prevediamo una condanna fino a cinque anni), e poi invece consentiamo che l'imprenditore o il cittadino che accettano il prezzo della corruzione ne siano esenti e non siano nemmeno chiamati alla denunzia. Ecco perché riteniamo che tutto vada riportato nell'ambito della corruzione e che l'ipotesi residuale della concussione per costrizione diventi invece un'ipotesi qualificata del reato di estorsione. L'altro punto qualificante è l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico di influenze illecite, espressamente contenuto nella Convenzione europea.

da chi fa credere, non da chi ha in effetti la possibilità di avvicinare i pubblici ufficiali ed i pubblici amministratori. Si intende pertanto introdurre nel nostro ordinamento

dietro pagamento, al servizio del richiedente per alterare la buona amministrazione avvicinando il pubblico ufficiale. Tale condotta non esiste nel nostro ordinamento, che prevede soltanto la condotta sanzionabile di chi millanti di poter fare questo senza invece averne la possibilità. Noi vogliamo che venga sanzionato chi ha tale possibilità, ossia le *lobby*, che sono una realtà pesante nel nostro Paese: ormai gestiscono loro i grandi affari. Riteniamo che questo

ordinamento. Altre previsioni normative consequenziali di minore livello, ma di uguale importanza sono l'inserimento del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per tutti coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione,

o per reati contro il patrimonio, qualora si tratti di truffe commesse in danno dello Stato o per la percezione di erogazioni da parte di enti comunitari o di usura. Riteniamo cioè che le persone che abbiano subito condanne per questi reati non possano continuare ad avere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, avendo

innanzitutto quella di rendere estremamente più facile la denuncia della corruzione,

infatti, chiediamo che innanzitutto venga unificato il reato di corruzione con quello di concussione per induzione. Badate bene che se c'è la concussione per induzione, cioè

Nel corso delle indagini di Mani pulite abbiamo visto che ogni volta che veniva incriminato qualche corruttore per corruzione tirava fuori la storia di essere stato indotto dal pubblico ufficiale e, quindi, che si trattava di una parte lesa. Dalle indagini poi risultava sempre che il cosiddetto concusso, che poi era un corruttore, aveva ricavato un grande vantaggio. Quindi, se noi vogliamo effettivamente che si scoprano di più la corruzione e la concussione, occorre che effettivamente il

Questo perché, signor Presidente, non c'è mai stato un caso di estorsione, che sia stato denunciato da chicchessia, che la polizia e la magistratura non siano riuscite a scoprire e ad arrestare in flagranza. Se noi effettivamente addiveniamo all'unificazione dei reati di corruzione e di concussione per induzione, così come del resto hanno suggerito anche i nostri rappresentanti internazionali

la cosiddetta legge ex Cirielli abbiamo notevolmente diminuito il termine di prescrizione. Se non adeguiamo le pene di questi nuovi reati unificati

concussione, tutto il giudizio, il dibattimento di primo grado ed anche in appello, si svolgono per stabilire se effettivamente si tratta della corruzione che è stata contestata o di concussione per induzione;

se ad un certo punto, in appello o anche addirittura in Cassazione, viene cambiata la qualificazione del reato, i reati naturalmente andranno in prescrizione, perché chi chi era parte lesa diventerà imputato, ma lo diventerà quando oramai è già quasi esaurito il processo o quando il suo reato di corruzione è già prescritto. Quindi, l'unificazione di questo reato, posto che alla fine dei conti viene punito il fatto che

per il reato permanente dal giorno in cui veniva a cessare la permanenza, ma il reato continuato venne eliminato, per cui si fece decorrere la prescrizione da ciascun reato consumato. Ora, quando si parla di corruzione che viene compiuta in continuazione, se facciamo decorrere la prescrizione dalla consumazione di ciascun reato, quando finalmente si riesce a scoprire un funzionario corrotto la maggior parte dei reati di corruzione

prescrivono tutti i reati commessi in precedenza, anche se il processo si riesce a svolgere velocemente. Pertanto, sebbene sia stato dichiarato inammissibile,

dopo aver estrapolato le norme dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale dai disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo. In Senato abbiamo già deliberato in ordine alla ratifica della Convenzione civile

Detto questo, gli emendamenti presentati dai senatori dei Gruppi del Partito Democratico e deall'Italia dei Valori sono molto simili nella impostazione di fondo, essendo basati innanzitutto sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale sia alla Convenzione di Strasburgo che alla Convenzione delle Nazioni Unite, in particolare nella ricomprensione della condotta di concussione per costrizione all'interno di quella di estorsione e della condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione, che impone la punizione tanto dell'erogatore quanto del ricevente somme di danaro o di utilità diverse per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario

del soggetto erogatore nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di millantato credito vantata anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato. non impiegato. Con entrambi i disegni di legge, e quindi con gli emendamenti presentati, si introducono circostanze attenuanti ad effetto speciale, con una diminuzione fino a due terzi applicabile alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari e anche al traffico di influenza in relazione alla persona che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi. Si introducono norme processuali idonee a potenziare i mezzi investigativi degli organi inquirenti con particolare riferimento all'agente provocatore. Si prevedono norme volte a sancire la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari. Inoltre, il disegno di legge già presentato a prima firma della senatrice Finocchiaro, e poi tradotto in emendamenti, prevede l'introduzione del delitto di corruzione privata, previsto dalla direttiva GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la cui attuazione era disposta dalla delega di cui alla legge comunitaria per il 2008, delega che non fu poi esercitata per la conclusione anticipata della scorsa legislatura. Si introduce una aggravante per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione relativa ai casi in cui il fatto sia commesso nell'ambito della gestione di calamità naturali o di grandi eventi. Si introduce l'articolo 319-*bis* del codice penale quale sanzione accessoria alla riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione. Si estende la confisca per l'equivalente di cui all'articolo Si tratta quindi di ridisegnare tutta la materia dei reati contro la pubblica amministrazione, innalzando sensibilmente le pene, che sono assolutamente inadeguate e che per determinati

sono soggetti ad una prescrizione molto più breve, dimezzata, oltre al fatto che vi è poi tutta una serie di strumenti che vengono indeboliti nella lotta contro la corruzione

l'esautoramento del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale in favore della polizia giudiziaria - è chiaro che queste norme sono assolutamente indispensabili perché si possa adeguare il nostro ordinamento, non solo alla Convenzione di Strasburgo, non solo alla Convenzione delle Nazioni Unite, che è legge dello Stato, ma soprattutto alla realtà dei fatti. In questo modo potremo finalmente cercare di spezzare quei rapporti tra pubblica amministrazione, malaffare, criminalità organizzata, politica e settore privato che purtroppo caratterizzano questi nostri tempi e che tutti, mi auguro, vogliamo evitare.

Signora Presidente, volevo intervenire su due emendamenti aggiuntivi che hanno a che fare in senso stretto con la lotta alla corruzione e con la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Dico subito che questi emendamenti sono stati dichiarati improponibili e che in precedenza, quando avevamo rilevato l'incomprensibilità

fa espresso riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. Sono le stesse Convenzioni internazionali - la Convenzione ONU del 2003 e la Convenzione di Strasburgo del 1999 - che ci parlano della necessità di una maggiore efficienza ed effettività nella lotta contro la pubblica amministrazione, dotando le forze di polizia e la magistratura di strumenti adeguati. Con questo emendamento si intendono sostanzialmente paragonare i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare quelli di corruzione e concussione, agli altri gravi delitti per i quali bastano sufficienti indizi di reato perché si possa procedere alle intercettazioni. Che si possa contestare il merito di una tale proposta emendativa è ovviamente comprensibile;

Gli altri due emendamenti sui quali vorrei soffermarmi, parimenti dichiarati improponibili - parimenti, a mio modo di vedere, in maniera incomprensibile - fanno riferimento alle modifiche dell'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione. Qui si tratta, nell'ambito contro la corruzione e per il massimo di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione, di fare in modo che i cittadini italiani siano messi a conoscenza dei fatti più gravi che si possono verificare nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai fatti di eccezionale rilevanza sociale. In questo senso, sono stati presentati gli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15 nei quali si fa esplicito riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Stati erano arrivati a condannare alcuni giornalisti per la pubblicazione di notizie coperte dalla riservatezza e che peraltro erano state ritenute di rilevante interesse sociale o addirittura di eccezionale rilevanza sociale. In quelle sentenze, ed in particolare in quella che ha condannato la Francia per avere a sua volta condannato i giornalisti, veniva scritto che la stampa i *mass media* sono come *le* *chien de garde*, il cane da guardia di una democrazia. Se noi eliminiamo la possibilità di controllo pubblico e di individuazione di questi reati, miniamo alla base un pilastro fondamentale della nostra democrazia. In questo senso, gli emendamenti che ho citato fanno esplicito riferimento alla trasparenza nell'attività di governo e della pubblica amministrazione e alla necessità di dotare gli organi investigativi degli strumenti necessari

(traffico di influenze illecite) e nello stesso tempo adeguare le pene sotto il profilo di un corretto rapporto con gli altri reati.

finestra"). Se non vi sono osservazioni, accantoniamo anche l'articolo 12. Onorevoli colleghi, è stato presentato dal Governo, ed è in distribuzione, l'emendamento 2.0.2000, in sostituzione dell'emendamento 2.0.1000

In questa maniera siamo assolutamente certi di quello che stiamo facendo.